non le ha poste; tanto meno ha messo in cima alla propria agenda politica il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Non ce n'è infatti traccia nei provvedimenti che sono stati affrontati e approvati in quasi sette mesi e mezzo:

Le soluzioni proposte dal decreto-legge in discussione non tengono conto di queste considerazioni e purtroppo fungono di nuovo da cerotto rispetto a un'emorragia in atto;

di regia non sono previsti in modalità definitiva e continuativa nemmeno gli enti territoriali preposti alla gestione della risorsa idrica, le autorità e gli istituti scientifici centrali e locali, che nelle audizioni hanno chiesto esplicitamente un coinvolgimento attivo e costante: una richiesta logica e fondamentale. Questo causerà seri cortocircuiti a livello locale e forti rallentamenti nell'applicazione del

che chiedono il potenziamento, la formazione e la riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche locali, per dare man forte nel sostenere, monitorare e avviare un'azione sostenibile, inclusiva,

si punta sull'efficiente gestione ordinaria della risorsa idrica e soprattutto alla corretta applicazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE e della direttiva alluvioni 2007/60/CE le due principali). È grave non prevedere la manutenzione delle reti di distribuzione delle acque a qualsiasi uso e non adoperarsi anche per la loro digitalizzazione, e ridurre ad esempio le perdite di acqua potabile che, in Italia, arrivano fino al 45

La convinzione diffusa è che, per fare presto, si devono bypassare procedure importanti per un territorio fragile come l'Italia, creando una giungla di eccezioni su eccezioni. Si pensa di semplificare e velocizzare, mentre invece si complica tutto ancora di più, compromettendo la realizzazione e la buona riuscita delle opere, allungandone paradossalmente i tempi.

quello di applicare deroghe su deroghe, che impattano su procedimenti e creano le basi per le scappatoie che di fatto danneggiano quel territorio e quell'ambiente che si devono poi andare a mettere in sicurezza quando il danno ormai è fatto.

Il risultato è deludente, dispiace prenderne atto. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra rinnoviamo l'appello al Governo di mettere in cima all'agenda politica il contrasto alla crisi climatica: mettete in sicurezza l'Italia e le persone che vi abitano.

genetica agraria, per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica ed in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità,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

La seduta è tolta